Onorevoli colleghi, un violento terremoto nella notte tra il 23 e il 24 agosto scorso ha 24 agosto scorso ha devastato alcune zone dell'Italia centrale colpendo, in particolare, le località di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto. L'Italia intera si è unita nel dolore, nel piangere l'impressionante numero di vittime e nell'ansia per la sorte dei feriti e delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Il triste bilancio di questa tragica calamità fa registrare ad oggi quasi 300 morti, tra cui numerosi bambini, circa 400 feriti ricoverati negli ospedali, più di 4.500 sfollati: numeri che compongono un quadro drammatico di esistenze precocemente interrotte, infanzie spezzate, famiglie lacerate, progetti e sogni di vita assurdamente svaniti, paesi e borghi travolti dalla forza devastante della natura. Oltre al pesante tributo di vite umane concorrono ad accrescere il nostro dolore i danni a un patrimonio storico, artistico, urbanistico di grande valore, parte importante della nostra identità e delle tradizioni culturali del Paese. Nel momento della tragedia e del dolore ha brillato lo straordinario e meritorio impegno degli operatori della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa, del Soccorso alpino, della Forze armate, delle Forze dell'ordine, delle strutture medico-ospedaliere e di tanti, tanti volontari. A tutti coloro che si stanno ancora oggi faticosamente prodigando nelle opere di soccorso e di assistenza vanno il plauso e la gratitudine profonda e sincera delle istituzioni e dell'intero popolo italiano. Essi rappresentano indubbiamente un esempio di quell'Italia migliore, capace di mobilitarsi di fronte alle emergenze, di accorrere in soccorso ai sofferenti, fornendo modelli ineguagliabili di abnegazione e spirito di fratellanza. È stata una vera e propria gara di solidarietà quella a cui si è assistito nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al sisma, con numerose persone in fila negli ospedali per donare il sangue o impegnate ad offrire spontaneamente sostegno e beni di prima necessità. Il più bel simbolo della rinascita dei territori colpiti si è avuto quando, questa mattina, è suonata la campanella per l'inizio del nuovo anno scolastico ad Amatrice. *(Applausi).* Tuttavia non può trascurarsi Tuttavia non può trascurarsi il parere degli esperti, secondo il quale un evento calamitoso di tale entità non avrebbe avuto effetti così drammatici in termini di vite umane e di devastazione se negli anni si fosse provveduto ad una più accorta programmazione nell'utilizzo del suolo e a una progettazione degli edifici pubblici e privati coscienziosa e rispettosa delle leggi esistenti. Certamente spetterà alle autorità competenti l'accertamento delle responsabilità connesse al mancato rispetto delle normative di appalto, di progettazione, di costruzione, di adeguamenti, con particolare riguardo agli edifici pubblici. Allo stesso tempo, tutte le istituzioni sono chiamate a concertare la propria azione per garantire che l'opera di ricostruzione si svolga nello scrupoloso rispetto delle vigenti norme antisismiche. Occorre, inoltre, dare risposta alle legittime e giustificate istanze sollevate dagli amministratori e dai cittadini coinvolti, affinché la ricostruzione tenda il più possibile al ripristino, graduale e sicuro, dell'originario tessuto urbanistico e delle comunità di appartenenza. Dobbiamo far rinascere i paesi colpiti perché costituiscono il punto di riferimento per la vita di tante persone, punto di riferimento che non deve essere cancellato, ma recuperato e trasmesso alle generazioni future, con la sua eredità di memorie e di tradizioni. Il Parlamento, in costante dialogo con il Governo e con le istituzioni territoriali interessate, sarà quindi chiamato, non solo ad adottare ogni misura di carattere legislativo funzionale alla ricostruzione, ma anche a monitorarne costantemente l'efficacia e la relativa tempistica di attuazione, a cominciare dalla predisposizione degli alloggi provvisori per le popolazioni sfollate e di tutte le infrastrutture necessarie per la ripresa delle attività economiche e sociali. Nel rinnovare quindi il cordoglio profondo del Senato della Repubblica per le vittime e nel formulare un sentimento di sincera vicinanza verso i feriti, le popolazioni sfollate e tutte le famiglie colpite, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

Componenti del Governo, ci troviamo purtroppo all'ennesima manifestazione di cordoglio nazionale. Non si vuole assolutamente strumentalizzare nulla: la tragedia è l'ultima di una lunga serie, ma ciò che è accaduto in passato, oltre a errori clamorosi, ci ha lasciato qualcosa di importante.

presenza del ministro Delrio per chiedergli di ripristinare innanzi tutto la viabilità. Il genio militare ha già dimostrato quello che sa fare.

Indirizziamo tutto il nostro impegno, l'impegno del Governo e di quest'Assemblea a far sì che questa gente seriamente abbia le risposte e che le abbia nei tempi più brevi possibili. Si può fare:

Questa è la prima esigenza. Quella gente chiede di stare a casa propria e nel più breve tempo possibile e bisogna creare le condizioni perché questo avvenga. Se questo non lo si farà

abbatterli o, se è possibile, ripristinarli in termini di serietà ed efficientismo antisismico. Non sono chiacchiere; è un'opera ciclopica che va fatta evitando ogni sorta di demagogia, perché se qualcuno vuole «infilarsi» per fare demagogia o fare *spot* elettorali di Governo o di minoranza, sbaglia. Sui problemi della gente, sui problemi dell'Italia non si gioca. Noi come Conservatori e Riformisti metteremo tutto il nostro impegno

sono i primi attori, insieme alla popolazione, rispetto a quello che deve accadere. È necessario che vengano coinvolti; devono poter dire la loro, non possono essere esclusi; devono essere i primi responsabili di quello che si fa e di quello che non si fa. Non accentriamo perché sbagliamo; accentriamo delegando, controlliamo, siamo «sul pezzo» attraverso tutte le nostre istituzioni, i nostri Ministeri, la Protezione civile. Controlliamo, ma non siamo ossessionanti, e liberiamoci da lacci e lacciuoli burocratici che bloccano spesso le opere e creano problematiche. Questa è la realtà. Diamo la libertà al cittadino di Amatrice che ha i mezzi finanziari di poter rinforzare e mettere a posto la casa senza aspettare che qualcuno gli dia l'autorizzazione; diamo le indicazioni su tutto il da fare. Questo ci aspettiamo: la fattività, la realtà. Le chiacchiere e le utopie se le porta il tempo. È il tempo delle risposte vere e immediate, abbiamo tutti i mezzi e le possibilità di farlo. Quanto alla generosità del popolo italiano, fino

I Vigili del fuoco, che non possono essere ancora così pochi, così malpagati e così male inquadrati (è il dato reale), hanno dato l'ennesima prova, come tutte le forze della Polizia e dei Carabinieri, di quanto siano affidabili per il Paese. Questo è il dato reale. Diamo risposte vere. Su questo aspettiamo il Governo, su questo aspettiamo l'intera Assemblea, perché è un problema che riguarda l'intera Assemblea. Non ci chiamiamo fuori: siamo i primi responsabili se non sappiamo controllare.

partecipa a questa commemorazione in ricordo delle vittime del terremoto che nella notte del 24 agosto ha colpito pesantemente il Centro Italia in quattro Regioni, in particolare nel Lazio e nelle Marche. Il bilancio del sisma è drammatico ed è di quasi 300 morti, tutti registrati in tre paesi: Amatrice (il più colpito), Accumoli e Arquata del Tronto. È un bilancio pesante, simile a quello del sisma dell'Aquila del 6 aprile del 2009, accaduto quasi alla stessa ora, quando persero la vita 309 persone. Il forte sisma ha anche inevitabilmente prodotto centinaia di feriti, la distruzione dei centri storici e di molte frazioni di questi tre paesi (fra tutti Pescara del Tronto, completamente rasa al suolo), la distruzione del patrimonio storico-culturale, oltre ad aver creato danni in altri centri dell'Umbria e dell'Abruzzo e conseguenze anche sul comparto economico, agricolo e del turismo in particolare. Alla data odierna sono quasi 4.000 le persone assistite soprattutto nei campi tenda e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi: quasi 1.000 nel Lazio, oltre 1.700 nelle Marche, 800 in Umbria e quasi 300 in Abruzzo. Con il collega Candiani alla fine di agosto ci siamo recati sui luoghi del sisma per capire la situazione e soprattutto le necessità di queste comunità. Abbiamo parlato con i cittadini, con i soccorritori e soprattutto con i tre sindaci che devono essere il perno della ricostruzione. Sui visi delle persone abbiamo trovato molta sofferenza, ma anche tanta dignità, voglia di ricominciare e di ricostruire la propria casa e il proprio ambiente. Per il *post* terremoto mi preme sottolineare come, a differenza del sisma dell'Aquila, in particolare sono due gli aspetti che destano preoccupazione: basse temperature che già si sono registrate, soprattutto di notte, nonostante l'inverno sia ancora distante, vista l'altitudine dei territori colpiti, e che metteranno a dura prova le genti assistite nei campi tenda; dato dalla distribuzione estesa delle zone terremotate, che presuppone una più impegnativa logistica per l'assistenza e la ricostruzione. Solo tra Amatrice, Accumoli e Arquata stiamo parlando di 100 frazioni su una superficie estesa di oltre 350 chilometri quadrati, ognuna con delle abitazioni dove i residenti colpiti vogliono - diciamo noi giustamente - permanere anche in tenda. Non ci dimentichiamo, inoltre, Il Gruppo parlamentare della Lega Nord rinnova i ringraziamenti a tutti coloro che dal primo istante si sono prodigati per assistere le popolazioni colpite: gli uomini della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, le donne e gli uomini del soccorso della Croce Rossa italiana quelli delle Forze dell'ordine, gli alpini, i tanti volontari che si sono resi disponibili per aiutare ad alleviare i problemi; le centinaia di tecnici, geometri e ingegneri che stanno correndo per verificare le condizioni statiche e di sicurezza delle case e degli edifici pubblici per l'agibilità. anche alla generosità di milioni di italiani che si sono mobilitati per la raccolta fondi e generi di prima necessità, rischiando persino di mandare in *tilt* la logistica. Ovviamente il Gruppo della Lega Nord esprime sentimenti di cordoglio a tutti i famigliari delle vittime e si stringe alle popolazioni colpite che hanno perso la propria casa, il proprio opificio, gli affetti. Il Gruppo della Lega Nord si augura che il Governo e il Parlamento varino senza indugio provvedimenti che possano rendere trasparenti, rapide ed efficaci le fasi del post-emergenza e della ricostruzione, con misure di fiscalità adeguate e con certezze economiche nei risarcimenti alle persone, alle famiglie e alle imprese che hanno perso tutto. Ovviamente seguirà anche il ragionamento sulla prevenzione. La Lega su questi punti sarà vigile, presenterà proposte serie e "marcherà stretto" il Governo. Non vogliamo speculazioni politiche e inutili passerelle di Ministri, che rischiano di essere una presa in giro, a danno di persone che hanno sofferto già troppo. *(Applausi dal

alla luce degli sforzi fatti affinché si realizzassero per tempo le opere necessarie a fare in modo che la scuola potesse riprendere anche per i ragazzi di quei Comuni, letteralmente devastati dal terremoto. Si tratta di un avvenimento molto importante, che ripaga anche degli sforzi fatti da tutti coloro che si sono adoperati per garantire che, anche ad Amatrice, le lezioni potessero oggi ripartire. Questo impegno e questa dedizione sono la rappresentazione di quello spirito che rende grande il nostro Paese e pronto a stringersi in maniera incondizionata attorno a chi ne ha bisogno. Lo si è visto,

in favore delle popolazioni colpite da questo evento catastrofico. Apprendere che i volontari intervenuti nelle aree colpite dal terremoto erano molti di più di quanti effettivamente occorressero è stato per me motivo di orgoglio e lo è stato per tutti gli italiani. Si tratta di un esempio di concreta solidarietà nazionale, che ha trovato la giusta dimensione anche nelle nostre istituzioni, che si sono univocamente mobilitate per dare quelle risposte certe e immediate, che era giusto fornire fin dal primo momento a quanti si sono ritrovati, nel giro di una notte, senza più nulla di quello che si erano costruiti negli anni. Tale coesione non ha lasciato spazi a strumentalizzazioni o a polemiche e ha certamente facilitato la messa in campo di misure concrete, per porre un freno alla situazione di emergenza più immediata. Adesso bisogna però archiviare definitivamente questa prima fase, per passare ad una successiva, che abbia i suoi effetti nel lungo periodo. È necessario accelerare i tempi il più possibile nel reperimento di quelle risorse necessarie non più esclusivamente ad affrontare la fase post-terremoto, bensì a superarla in maniera più o meno definitiva. Insistere sulla richiesta rivolta all'Europa di una maggiore flessibilità per far fronte all'emergenza in maniera adeguata è certamente un primo importante passo. Quello stesso spirito, che ha animato gli italiani, dovrebbe spingere alla solidarietà e alla coesione anche gli altri Paesi dell'Unione. Sarebbe un grande e concreto esempio di quello "spirito europeista", di cui tanto si parla, ma che troppo spesso stenta a palesarsi nella quotidianità. C'è poi un altro aspetto che deve essere posto in primo piano, sempre in un'ottica squisitamente costruttiva e non polemica: quello della prevenzione. Molti centri storici dei Comuni italiani sono a rischio sismico. Si tratta di aree che appartengono al nostro patrimonio culturale, che va sicuramente salvaguardato, il che rende, ad esempio, ingeneroso un paragone con il Giappone e con le infrastrutture antisismiche lì realizzate. Bisogna però, al contempo, mettere in sicurezza questi centri a rischio, pur salvaguardandone la valenza storica. Si pensi ad esempio alla Turchia, dove per far fronte alle pessime condizioni di un patrimonio abitativo mal ridotto, si sono temporaneamente collocati presso abitazioni prese in affitto gli abitanti delle case che necessitano di interventi di messa a norma. È necessario cominciare subito con un piano di messa in sicurezza degli edifici a rischio anche in Italia. Non si tratta di un'operazione facile, ma va comunque certamente organizzata in tempi rapidi, perché sul tavolo c'è l'incolumità degli italiani. E questo è tanto più vero se pensiamo agli edifici pubblici e alle scuole o alle strutture ricettive di un pubblico molto giovane in particolar modo. La sicurezza è per i cittadini un diritto, cui lo Stato ha il dovere di ottemperare. L'auspicio del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie è dunque quello che, già nel corso dei lavori sulla legge di stabilità, così come si era da più parti convenuto, si individuino effettivamente gli interventi più urgenti da effettuare e le risorse necessarie alla loro attuazione. Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, a nome del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE, esprimo la nostra solidarietà per la tragedia che ha riguardato le comunità del centro Italia, una tragedia che ha generato un dolore per le persone che non ci sono più, per quelle che oggi piangono i loro cari e che devono trovare la forza per rialzarsi e per ritornare a vivere. È in situazioni del genere che le istituzioni e tutto il Paese devono dare il meglio di sé. Troppe volte nella storia repubblicana, attorno a tragedie tanto gravi, si è unita la vergogna: vergogna per chi ha speculato o ritardato i lavori, per gli sprechi, per gli appalti gonfiati, per la scia di malcostume e corruzione che hanno generato. Per fortuna non è sempre stato così. Ci sono state anche pagine importanti, in cui le istituzioni e la politica in generale hanno dato prova di grande responsabilità, di abnegazione e di spirito di servizio. Oggi i cittadini di Amatrice e degli altri Comuni colpiti dal terremoto, tutte le italiane e gli italiani guardano con attenzione al modo con cui le istituzioni sapranno operare per la ricostruzione, per dare nell'immediato condizioni di vita accettabili, per riallacciare i nodi del tessuto sociale e di quello economico. E lo fanno con gli occhi di chi, in queste settimane, ha scritto pagine commoventi di profonda solidarietà e vicinanza, attraverso le raccolte fondi, l'invio di generi di prima necessità, il lavoro sul territorio delle reti di volontariato e delle squadre della Protezione civile di tutta Italia,

i bambini di Amatrice possono iniziare l'anno scolastico grazie ai prefabbricati costruiti dalla Provincia autonoma di Trento, che questa mattina sono stati inaugurati dal ministro Giannini e dal presidente della Provincia Ugo Rossi, che per l'occasione ha portato ai bambini di Amatrice i disegni e i regali dei bambini del Trentino. La nostra Protezione civile è stata tra le prime ad accorrere per prestare soccorso ai sopravvissuti e contribuire alle operazioni di recupero dei corpi delle vittime. Voglio ringraziare tutti gli operatori e i volontari, qui in quest'Aula, così come ringrazio, a nome di tutti i trentini, tutti quelli che in queste settimane hanno raccontato di un Paese che, nei momenti difficili, sa compattarsi in un solo secondo intorno ai valori della solidarietà, dell'amicizia e della fratellanza. La velocità con cui è stato possibile l'intervento del Trentino, sia nella ricostruzione della scuola, sia nell'attivazione della Protezione civile, per giungere all'immediata attivazione del fondo di solidarietà per raccogliere nuove risorse per specifici progetti di ricostruzione, gestiti direttamente dalla Provincia, permette anche di capire cos'è la nostra autonomia: una terra solidale come tantissime altre, certamente, ma soprattutto un modello di governo che permette alla comunità di poter esprimere al meglio questa sua vocazione, che continuerà a fare la sua parte, così come è chiamato a farla anche il Governo nazionale. Siamo d'accordo con il presidente Renzi sulla necessità di un piano straordinario attorno al quale si ritrovino tutte le forze politiche e sociali, senza distinzione alcuna. Accanto a queste risorse, decisivi appaiono gli incentivi ai soggetti e agli investimenti privati. In questa prospettiva, hanno un ruolo fondamentale sia le misure di semplificazione che il rafforzamento e l'allargamento degli incentivi fiscali, che siano aggiuntivi ad esempio agli *ecobonus*, adeguati agli obiettivi di ristrutturazione antisismica. I dati relativi all'azione e alle misure di prevenzione antisismica sono un punto strutturale e dirimente, se pensiamo che i benefici sono stimati in una media pari ad un risparmio di quattro euro di costi per la ricostruzione per ogni euro investito nella prevenzione; incentivi che siano flessibili e dunque differenziati in relazione a diverse tipologie e che impongono in primo luogo un serio censimento delle situazioni a rischio e con la priorità attribuita alla messa in sicurezza di scuole e ospedali. Ruolo centrale dovrà essere dato ai sindaci delle comunità interessate, nella definizione di un piano organico di intervento, con l'idea che non si debbano costruire *new town* (modello applicato all'Aquila e rivelatosi del tutto errato), ma attraverso cantieri leggeri, entro un quadro di coordinamento, un sistema di cooperazione pubblico-privato fondato su crediti fiscali, con un ruolo fondamentale della Cassa depositi e prestiti e una valutazione dei costi affidata agli enti locali, già sperimentata in Emilia Romagna, e con un ruolo centrale dell'Autorità di vigilanza anticorruzione. Condividiamo quanto espresso dal senatore a vita e collega del nostro Gruppo, Renzo Piano, in merito al senso complessivo degli interventi. Occorre essere consapevoli di dover adottare politiche che interesseranno le prossime generazioni e nelle quali l'attuale fase di emergenza sia concepita come un problema...

partecipiamo oggi commossi, come senatori di Sinistra italiana e del Gruppo Misto, alla commemorazione di 296 persone, donne, uomini e bambini, che venti giorni fa hanno perso la vita sotto le macerie delle loro case, abbattute dal terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto ha colpito Amatrice, Accumoli, Arquata, Pescara del Tronto e molte aree limitrofe nell'Italia centrale.

nelle prime ore dopo il terremoto, affidando la nostra solidarietà, non solo a parole e a messaggi, pur sinceri, ma anche a gesti concreti.

la solidarietà espressa da milioni di italiani, subito, nelle prime ore dopo la tragedia. Si dice che i terremoti non possono essere previsti, ma dobbiamo dire che questo è vero solo in parte. Non si possono prevedere il giorno, l'ora e il luogo preciso, ma sono note a tutti noi le zone a maggior rischio, quelle dove sarebbe stato necessario e urgente intervenire preventivamente. L'area colpita il 24 agosto era una di quelle ad altissimo rischio sismico, sulla quale si sarebbe intervenire per porle al riparo senza attendere che si verificasse la tragedia. Ma non è stato così, come per moltissime altre parti dell'Italia. Si dice che dalle catastrofi naturali non ci si può difendere, ma anche questo è vero solo in parte: anzi, in minima parte. In altre zone del mondo ad alto rischio sismico sappiamo che gli edifici hanno resistito e che sono in grado di resistere. Certo, il nostro territorio e i nostri borghi sono diversi per complessità urbanistica e per storia. Ma era possibile, anzi sarebbe stato doveroso (e vedremo ora come si ricostruirà) intervenire in modo diverso. Non dobbiamo ignorare, perché altrimenti non diciamo le cose come stanno,

di pietra ricoperte di tetti di cemento armato. Tutto questo è accaduto e tutto questo è quanto noi dovremo tener presente per affrontare l'opera della ricostruzione. Oggi l'urgenza prioritaria e assoluta è dare il prima possibile un tetto agli sfollati. I sette mesi previsti - lo abbiamo detto e lo ripetiamo - ci sembrano un tempo troppo lungo; forse si può abbreviare, soprattutto alle soglie dell'inverno. Occorre fare presto e avviare immediatamente il piano per la ricostruzione. Con altrettanta chiarezza abbiamo avanzato le nostre proposte: deve continuare il confronto su come avviare l'opera di ricostruzione. Abbiamo avanzato una proposta precisa: l'allocazione, ad esempio, di metà del fondo per le esigenze indifferibili in capo alla Presidenza del Consiglio per affrontare l'emergenza nelle aree terremotate e avviare immediatamente un'opera seria di ricostruzione. Non possiamo più accontentarci di interventi *ex post*. Troppe volte ci siamo trovati a dover commemorare le vittime di qualche sciagura e di qualche tragedia. Troppe volte ci siamo ripetuti che si sarebbe potuto, se non evitarle, almeno minimizzarne le conseguenze. È ora di farlo davvero, è ora di attuare una vera e propria rivoluzione copernicana: cambiare profondamente l'impianto culturale e progettuale e avviare - vedo qui il ministro Delrio - un grande piano per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, un piano certamente decennale, basato su interventi pubblici, detrazioni fiscali, nuove tecnologie, formazione degli operatori, che preveda non solo la ristrutturazione delle case e degli edifici, ma anche la messa in sicurezza del nostro territorio. Ricordo che in Italia il 60 per cento degli edifici risale a prima dell'entrata in vigore delle norme sulla sicurezza del 1974 e anche quelle costruite dopo hanno spesso ignorato queste norme, come purtroppo molti casi di edifici colpiti dal terremoto confermano tragicamente. Oggi è il giorno della tristezza, del cordoglio per i morti e della solidarietà ai feriti e agli sfollati ma deve essere - Presidente, lo dico a tutti noi e al Governo - anche il giorno della serietà e degli impegni precisi se non vogliamo trovarci, in un prossimo futuro, di nuovo qui a piangere altri morti e davanti ad altre tragedie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'ennesima tragedia e i momenti di dolore che hanno colpito il popolo italiano, i numerosi appelli alla comune responsabilità necessitano di risposte concrete ed immediate. Tutto il Paese si è stretto in un grande abbraccio di solidarietà attorno alle popolazioni colpite. La società tutta e la macchina dei soccorsi, come sempre, hanno risposto in modo egregio mobilitando risorse umane, strumentali ed economiche che solo popoli generosi come quello italiano riescono a garantire. Ne approfitto pertanto per ringraziare le autorità locali, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze di polizia e il Corpo di polizia di Roma Capitale, le Forze armate e i volontari, per l'impegno e la dedizione manifestata nell'opera di soccorso, ciascuno con ruoli e compiti differenti ma tutti animati da un sincero spirito solidale e comunitario. Ora tocca alle istituzioni dare la risposta più importante. La risposta sarà davvero efficace se si porrà al centro di qualsiasi progetto o campagna la parola «prevenzione». Ma che non sia più una parola usata per *spot* estemporanei e poi richiusa in un cassetto. Prevenzione vuol dire investire soldi, molti purtroppo per il ritardo accumulato dal nostro Paese, per garantire un reale adeguamento antisismico delle opere edilizie, *in primis* di quelle che si trovano nelle fasce territoriali a più elevato rischio La prevenzione necessita di una mappatura certosina degli edifici esistenti in modo tale da costruire un fascicolo del fabbricato, una sorta di carta d'identità dell'edificio. Sono oltre 900.000 i fabbricati abitativi che si trovano nelle aree di massimo rischio e circa 93 miliardi è il costo stimato. Fino ad oggi si è puntato sull'adeguamento sismico volontario attraverso la detrazione del 65 per i lavori di antisismica, per il momento in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le prime case e gli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. signor Ministro, certamente utile, dovrà essere rafforzata ed estesa, ma non potrà rimanere l'unica azione messa in campo come risposta ad anni di ritardo. Dobbiamo fornire una risposta seria ed adeguata e non lo dobbiamo solo alle vittime di Amatrice e del Centro Italia, ma a tutte le vittime dei passati eventi calamitosi, dal Belice all'Irpinia, dall'Umbria all'Aquila e all'Emilia, a tutti coloro che dopo eventi del genere non solo hanno perso dei cari ma hanno visto le loro abitazioni e i loro paesi cadere in pezzi; territori e popolazioni che oggi, anche a 48 anni di distanza, signor Ministro, aspettano una risposta e la chiusura di questa drammatica parentesi del loro vissuto. tanto quanto la prevenzione, è ora la fase di ricostruzione: le istituzioni coinvolte in questo lungo e complicato processo si devono adoperare affinché sia seria e tutti i centri colpiti tornino a vedere la luce lì dove sono sprofondati. Solo così la forza di queste comunità silenziose non verrà dispersa, solo così un giorno le campane potranno ritornare a suonare a festa. Simbolo della ricostruzione può essere la scuola elementare di Amatrice: la Protezione civile di Trento ha costruito in tempo *record* un edificio modulare che ha consentito a più di duecento bambini di iniziare puntualmente l'anno scolastico. Ora dovranno ricevere simile attenzione anche tutti quegli scolari che negli altri paesi saranno costretti a tornare alle lezioni in prefabbricati, tende e strutture attrezzate. L'attenzione e la vicinanza alle popolazioni nel lungo periodo sarà uno dei fattori decisivi per la rinascita. I riflettori non dovranno accendersi solo in occasione delle visite istituzionali, ma dovranno garantire l'informazione puntuale e la stretta vigilanza sullo svolgimento delle fasi della ricostruzione. A livello centrale, il Parlamento, in accordo con il Governo, deve immaginare misure e strumenti affinché tali tragedie non si ripetano più: serve lo stanziamento di risorse importanti, da utilizzare secondo criteri efficaci e con la supervisione coordinata di strutture locali e centrali. La magistratura procederà anche con tutti gli accertamenti opportuni per verificare che nel passato siano stati rispettati i parametri nella costruzione degli edifici pubblici. Già oggi sul territorio opera il commissario per la il commissario deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare con mezzi rapidi, in accordo con i rappresentanti delle istituzioni locali e senza essere ostacolato dai cavilli della burocrazia. se ciascuno dedicherà ogni energia al compito ricevuto, il lavoro di squadra potrà riconsegnare alle popolazioni colpite una nuova normalità e potremo dire di aver onorato la memoria di tutti i caduti in questa terribile calamità e in quelle che l'hanno preceduta.

nel 1976 in Friuli, con 990 vittime; nel 1980 in Irpinia, con 2.914 vittime; nel 2002 a San Giuliano di Puglia (lo ricordiamo tutti, con una classe sepolta); nel 2009 a L'Aquila, con 309 vittime, e 20 e 29 maggio 2012 in Emilia con 27 vittime. Questo triste, ma triste, elenco avrebbe dovuto insegnare qualcosa, gestione dell'emergenza, ma anche nella prevenzione e riduzione degli effetti dei terremoti. Invece è arrivato il 24 agosto, il Centro Italia ha tremato, con 296 vittime e migliaia di sfollati. Le nostre istituzioni hanno puntato sull'emergenza e per la prima volta in Italia si è vista una buona organizzazione: gli arrivi di mezzi ed uomini sono stati immediati e a questi spetta la nostra infinita riconoscenza. La loro efficienza e competenza è testimoniata dal numero delle persone estratte vive da quei cumuli di macerie, davvero impressionanti. Ma il terremoto ha fatto emergere anche situazioni imbarazzanti; molti edifici pubblici, come la scuola e l'ospedale di Amatrice, appena ristrutturati, non hanno resistito alle scosse, evidenziando come l'ingordigia e l'interesse personale abbiano prevaricato sull'interesse per il bene pubblico. Spero che la ricostruzione non racconti mai più fatti come quello del Comune di Fossalto. Per chi non lo sapesse, questo piccolo Comune di 1.400 anime del Molise è stato colpito dal terremoto di San Giuliano di Puglia. La scuola aveva superato brillantemente il terremoto, con qualche piccola crepa sull'intonaco, ma si è deciso di aumentarne la resistenza, spendendo 473.000 euro. Dopo due anni di uso, con tanto di feste, le insegnanti chiedono le certificazioni antisismiche, che non sono mai arrivate. Vengono chiamati i consulenti e si scopre che la scuola non è più agibile e ora, per portarla allo stato di agibilità, ci vuole più di un milione di euro. Concludo ribadendo che molte delle vittime del terremoto del 24 agosto scorso potevano essere evitate, se solo si fosse costruito in modo diverso, se fossero state date le giuste informazioni, privilegiando il principio del bene comune. Invece siamo qui a ricordare tante vittime e farci carico dei superstiti, che hanno perso non solo la casa e i loro effetti personali, ma molto spesso anche i loro cari e anche il senso di comunità. Mi auguro che la vicinanza che annunciamo con tanta enfasi in questa Aula sia testimoniata da provvedimenti legislativi che consentano loro un ritorno ad una vita normale in tempi brevi. E mi sento, infine, in dovere di ricordare che il Movimento 5 Stelle auspica da sempre provvedimenti per la messa in sicurezza dell'Italia intera, onde evitare simili tragedie. *(Applausi

schierate in quella palestra con i familiari accanto provati dal dolore. Un ringraziamento particolare credo lo dobbiamo alla Protezione civile, ai volontari che si sono spesi in tutti i modi e alle Forze dell'ordine, che hanno salvato più di 60 persone dalle macerie.

a me preme far comprendere al Senato quanto questo terremoto abbia dimensioni più gravi rispetto a quanto si possa immaginare.

il Parlamento deve dare una risposta adeguata. Servono procedure semplici; non ci complichiamo la vita. Ho partecipato ad alcune riunioni e sono rimasto basito nel sentire che i sindaci dovrebbero chiedere alla Protezione civile il legname per fare una balaustra per mettere in sicurezza una struttura. Siamo al ridicolo. Ogni sindaco,

dando priorità assoluta all'Appennino centrale, dove i sismi si ripetono con continuità. Durante il dibattito parlamentare le opposizioni pretesero che la funzione non venisse assegnata alla Protezione civile, ma alle Regioni. A distanza di otto anni, nulla è stato fatto in questo senso, anche il parere della Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni però non hanno ottemperato a questo obbligo. Mi pare che molto sia da fare in questo senso. Errani era il presidente di quella Conferenza Stato-Regioni, quindi forse

Signor Presidente, le senatrici e i senatori del Partito Democratico, nel ricordare il dolore della notte del 24 agosto, abbracciano chi ha perso i suoi cari, sono vicini ai feriti e solidali con chi è stato colpito nei beni personali o ha visto distrutti i beni comuni della sua comunità. Il terremoto ha lasciato centinaia di morti e tantissimi feriti, ha raso al suolo interi Comuni, ha colpito duramente l'economia di un vasto territorio dell'Appennino centrale, ha abbattuto migliaia di case del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria. Hanno ragione i cittadini a non voler abbandonare i luoghi dove hanno sempre vissuto e a volerci tornare dopo la ricostruzione. Il Parlamento deve comprendere i sentimenti profondi che legano quelle popolazioni alle proprie terre e difendere abitudini e stili di vita fondati su culture antiche e tradizioni di grande valore. Molta gratitudine va a chi ha onorato l'Italia in operazioni di soccorso, difficili e rischiose, arrivando immediatamente sui luoghi del sisma e rimanendovi sino a quando c'è stato bisogno: donne e uomini della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e delle Forze armate, del soccorso alpino e speleologico, tanto personale civile dello Stato, delle Regioni e dei Comuni e moltissimi volontari è stata straordinaria, e dobbiamo darne atto, la generosità di decine di migliaia di italiane ed italiani che stanno aiutando con donazioni in denaro i paesi colpiti dal terremoto. Abbiamo visto in televisione le facce di soccorritori di tutte le età, segnati dalla stanchezza ma mai rassegnati, pallidi per la fatica; facce sporche di sudore e di polvere, con gli occhi febbrili per l'ansia e la tensione. Abbiamo visto visi di persone generose, che hanno mostrato competenza e professionalità sapendo che da ogni loro passo, da ogni loro movimento, da ogni loro decisione anche minima dipendeva la vita o la morte di donne, uomini e bambini. Abbiamo visto le qualità migliori degli italiani migliori. Guardando quelle facce, abbiamo sentito l'orgoglio di essere italiani. È stato detto che la responsabilità di tante morti dev'essere attribuita non al terremoto, ma alle azioni scorrette dell'uomo. Non so e non credo che oggi qualcuno possa distinguere con sicurezza tra gli effetti del terremoto e le responsabilità per i comportamenti e per le omissioni umane. Ma sappiamo che le famiglie, i sopravvissuti e l'Italia l'Italia intera hanno diritto alla verità e che nel nostro ordinamento la magistratura ha il compito di farcela conoscere. Lasciamo che sia la magistratura a lavorare con equilibrio e giustizia ed impariamo ad aspettare le sue conclusioni, senza cercare di anticiparle con le nostre supposizioni o, peggio, con le nostre aspirazioni politiche. Ancora poche parole sul futuro. La ricostruzione sarà un'impresa difficile e molto lunga, ma andrà bene. Il Governo è stato presente nei territori colpiti fin dal primo istante con il ministro Delrio; il commissario Errani è un galantuomo ed è persona molto

Dobbiamo guardare avanti, al futuro dei territori colpiti e delle città devastate, ma dobbiamo anche ricordarci che dal passato c'è sempre molto da imparare, non solo nel bene - e penso da ultimo al Friuli, all'Umbria e all'Emilia-Romagna ma anche per non ripetere errori già fatti, specie nella scarsa vigilanza e nello spreco di risorse. Oggi l'Italia è chiamata ad andare oltre le sfide del soccorso immediato e di una responsabile ricostruzione. Il Governo italiano si è posto l'obiettivo ambizioso e di lungo termine della messa in sicurezza del nostro patrimonio storico, monumentale, abitativo e paesaggistico. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia le nostre responsabilità e riconoscere la profondità del ritardo nella prevenzione del rischio sismico. Non tutti i pericoli derivanti da fenomeni naturali possono essere previsti e neutralizzati, ma le nuove conoscenze scientifiche, l'esperienza e una buona prevenzione possono ridurne al minimo gli effetti negativi. Molte volte, dopo i terremoti abbiamo affrontato la costosa e difficile attività di ricostruzione di città e territori distrutti. L'Italia è considerata un'eccellenza per la capacità ampiamente dimostrata nella gestione delle emergenze, ma siamo davvero molto indietro nella prevenzione e nella manutenzione. In passato Governi di ogni colore hanno saputo affrontare le calamità naturali, ma nessun Governo, né di destra né di sinistra, ha mai avuto la lungimiranza di avviare un programma serio e di lungo periodo per mettere in sicurezza le parti più deboli del nostro Paese. Nessuna forza parlamentare, pur avendone gli strumenti, ha incalzato i Governi con l'insistenza necessaria perché si muovessero, né mai c'è stata quella pressione continua e ripetuta dei *media* e dell'opinione pubblica che su altre questioni ha spesso mostrato di saper produrre risultati positivi. Oggi sappiamo che è possibile fare prevenzione

per i quali la sicurezza statica è indispensabile quanto la tutela dei loro valori artistici. Di grande importanza per il futuro del nostro Paese che il programma di messa in sicurezza dell'Italia sia stato assunto come prioritario dal Governo, così come è indispensabile che, con altrettanta priorità, venga sollecitato un coinvolgimento dell'Europa, il cui contributo non dovrà mancare. Questo

aiutare il nostro Paese a mettere il suo territorio al riparo, per quanto possibile, dai pericoli dei terremoti e dalle conseguenze delle nostre fragilità idrogeologiche. Per non cadere nella retorica, per non fare soltanto vuoti discorsi parlamentari, questo dovere deve essere da oggi l'impegno solenne del Senato. Signor Presidente, signori senatori, vi ringrazio innanzitutto perché credo che l'abbraccio che il Parlamento, insieme al Governo, ha voluto dare oggi, ricordando le 295 vittime del terremoto del 24 agosto, alle ore permette in qualche modo ai centri colpiti, alle popolazioni, alle famiglie, di sentire vicina la nostra Repubblica, tutta insieme, nelle sue articolazioni. Il primo pensiero doveroso va a queste vite interrotte, tra cui ben 22 minori: un dolore e una perdita che niente potrà colmare, ma che impegna tutti, come è stato e come continuerà a essere, a essere presenti, a essere tenacemente vicini ogni giorno, per restituire il più possibile una vita normale a chi ha subito un così grande dolore. Noi siamo lì, siamo stati lì fin dal primo momento, a nome del Governo ma credo anche a nome vostro, con la compassione e con la voglia di reagire e di andare avanti con determinazione,

lo ha fatto in tutte le sue componenti, cioè con i Vigili del fuoco, la Croce Rossa italiana, le Forze armate (questo è il Sistema della protezione civile) e le protezioni civili regionali.

alle ore 5 del pomeriggio e chiedere scusa perché volevano mangiare qualcosa. Ci hanno chiesto scusa: scusateci, mangiamo qualcosa, sono 10-12 ore che lavoriamo. Questa è un'Italia indimenticabile. Credo che il plauso al Sistema di protezione civile vada, appunto, anche alle Protezioni civili regionali che hanno dimostrato prontezza: è stato già citato il fatto che la Protezione civile del Trentino ha allestito da oggi la scuola e quindi l'anno scolastico è cominciato anche per i bambini di Amatrice. Avevamo detto fin dall'inizio che la ripresa delle attività scolastiche era un segno importantissimo,

Sappiamo che la normalità non è solo il primo giorno di scuola, ma il fatto di restituire anche la possibilità del lavoro. Per questo la Protezione civile, non solo sta compiendo tutte le

da ex sindaco di un Comune terremotato, ricordo la determinazione degli imprenditori della mia terra che dicevano di voler subito ricominciare a lavorare. Il lavoro, la scuola, la ricostruzione del Comune, del municipio, inteso come la casa di tutti: questi sono gli obiettivi che ci siamo dati

ma bellissimi centri della dorsale appenninica vadano ricostruiti, perché l'Italia è quella. In questo senso credo che il Governo abbia già fatto dei passi importanti prima di questa tragedia, come il piano per l'edilizia scolastica e il piano per la prevenzione del dissesto idrogeologico; inoltre ha già messo a disposizione le risorse per la ricostruzione per la prima volta grazie alla vostra azione si avrà di nuovo l'approvazione della nuova legge sulla Protezione civile. Per questo il Governo ha affermato di essere pronto a dare tutto il sostegno necessario perché la ricostruzione avvenga e avvenga lì; esprimevamo questa fortissima determinazione, abbiamo anche detto a tutto il Paese di aiutarci: è un'opera troppo difficile, abbiamo bisogno delle migliori intelligenze, dei nostri straordinari ingegneri, degli architetti. La disponibilità del professor Azzone e di Renzo Piano per citare i due più famosi, non deve però nascondere la grandissima disponibilità che abbiamo trovato da tutti i professionisti, le persone più comuni, per dare una mano a fare in modo che la ricostruzione sia vera, sia armonica, sia rispettosa

predisporre un inverno non troppo difficile per le popolazioni colpite, ma abbiamo già pronti tutti gli alloggi e le disponibilità per togliere le tende prima possibile. La vera sfida è quella di allestire le casette temporanee nel più breve tempo possibile e certamente cercheremo di fare ancora prima di sette mesi: abbiamo già individuato le aree e stiamo già ragionando su come accelerare le opere di urbanizzazione.

cura, manutenzione, prevenzione per il territorio e per i nostri luoghi pubblici. Le nostre scuole, le nostre piazze, le nostre chiese, i nostri ospedali sono il patrimonio della nostra identità: dobbiamo impedire che le nostre scuole o i nostri ospedali crollino, come purtroppo è successo ad Amatrice e nei luoghi colpiti dal sisma. Questo è il nostro obiettivo: realizzare un piano serio e credibile di prevenzione, che abbia delle priorità

tempo. Ciò che i nostri cittadini ci chiedono e chiedono a voi, oggi - e vi ringrazio per averlo manifestato così apertamente - è di essere con loro giorno dopo giorno,

di una comunità più forte, che potrà abbandonare i riflettori, ma non certo per essere dimenticata. Si spegneranno le luci e i riflettori, ma dobbiamo continuare a ricordare

passiamo ad esaminare l'articolo 2, in cui si ridefinisce la disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Nell'articolo 2 si definiscono i soggetti che potranno beneficiare di questi contributi e, giustamente, al punto 2) 2 si escludono «tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati», proprio perché si vogliono destinare i fondi a soggetti che svolgono veramente l'attività di informazione. Mi sono reso conto che, durante l'esame in Commissione, ci siamo dimenticati di uno dei requisiti che credo debbano essere basilari rispetto al fatto di poter beneficiare di questi contributi: coloro che beneficiano di questi contributi non possono avere

verrebbero nel caso usati per pagare degli stipendi, all'interno di questi giornali, che superano il tetto dei 240.000 euro. Quindi con il mio emendamento si fissa

alcuni emendamenti per noi assolutamente fondamentali sono già stati accolti in Commissione; quindi su questo non torno. Vorrei soltanto porre all'attenzione del relatore e dell'Assemblea

pubblici e trasparenti la partecipazione societaria dei giornali e delle imprese editoriali, il loro stato patrimoniale, le trasformazioni e gli aggiornamenti. Credo che questo

Ci sono anche altre questioni, che abbiamo sottolineato con la presentazione

desidero segnalare al relatore l'emendamento che riguarda il tema dell'attività editoriale

come questo aspetto possa essere sciolto all'interno del testo e, quindi, chiedo, eventualmente, di valutare una possibile riformulazione.

Le riviste scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di contributi volontaristici e molte di esse sono state già costrette a cessare le pubblicazioni. Si tratta di una perdita secca per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale con questa legge si potrebbe ovviare, peraltro con risorse molto limitate. Pertanto, invito il relatore a valutare l'opportunità di reinserire anche le riviste scientifiche fra i soggetti

L'espressione è palesemente vaga, e anche un po' ambigua, e non corrisponde all'esigenza, di cui molte aziende e cooperative editoriali hanno reso conto durante le audizioni in 1a Commissione,

sua cattiva qualità - sono spesso dovute, in questo Paese, non solo al controllo diretto che partiti e *lobby*, con enormi conflitti di interessi, esercitano direttamente sugli organi di informazione, ma anche al ricatto del precariato, come già è stato fatto

Nel testo licenziato dalla Commissione è scritto: «garantendo la massima rappresentatività territoriale». È evidente che si tratta di un'indicazione opportuna. le seguenti: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in proporzione al numero degli iscritti ed in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni Regione».

maggiore visibilità e vogliono raccogliere consenso in tutta Italia. Questo renderebbe il Consiglio dell'Ordine massimamente rappresentativo e ci garantirebbe un elemento di democraticità importante.

conformemente a quanto già stabilito in sede referente, nonché le proposte 2.128 e 2.175. Invito il

parere favorevole con una diversa formulazione: anziché sopprimere la parola «unicamente», introdurre, dopo le parole «imprese editrici che,», le parole «in ambito commerciale», in modo da specificare che l'attività che deve essere esercitata esclusivamente è quella in ambito commerciale.

se siamo al 77° posto per libertà di stampa nel mondo, dietro al Botswana, è grazie anche alle sovvenzioni dirette e indirette e all'occupazione militare dell'informazione, che vede poco pluralismo e molto clientelismo e sudditanza. Nel settore dell'informazione praticamente non esistono editori puri, non sono stati risolti i conflitti di interesse, non si fa niente contro le querele temerarie e vige il problema dell'intimidazione della mafia e della 'ndrangheta. Sono, infatti, tra i 30 e i 50 i giornalisti sotto protezione perché minacciati. Qui si sta parlando delle ricche elemosine di Stato che hanno trasformato questa editoria in un'editoria di Stato (1,5 miliardi in dodici anni).

modificano con una manina il contenuto, sapendo benissimo che il titolo incide più di quanto scritto in seguito, e ciò avviene anche perché la stampa risponde

Noi abbiamo combattuto una battaglia su questo, fin dal cosiddetto V-day del 2008, quando abbiamo raccolto 1.350.000 firme in un solo giorno per la libertà di stampa. sulla libertà di stampa e sull'abolizione del contributo all'editoria abbiamo presentato un disegno di legge che è stato il primo esperimento di democrazia diretta *online*: migliaia di cittadini sono intervenuti per dire che andavano abrogate tutte le disposizioni che prevedevano finanziamenti all'editoria, tranne quelle

OPA ostile all'interno del partito per conquistare la segreteria. Diceva che avrebbe tolto quei soldi ai giornali per darli agli asili nido. E adesso cos'è cambiato? Perché Matteo Renzi è passato dall'abolizione dei finanziamenti al desiderio di gestirli? Probabilmente serve una cassa di risonanza in piena campagna referendaria; serve a dare al Governo un potere di condizionamento sull'editoria attraverso una legge delega che permetterà di stabilire con quali criteri questo e quello dovranno prendere finanziamenti pubblici, e cioè soldi degli italiani, per falsare l'informazione durante la campagna referendaria. Noi non possiamo accettare questo. È una battaglia di libertà e coerenza che dovrebbe investire il Governo per il diritto dei cittadini a essere liberi e informati nel momento in cui devono votare. Abbiamo visto vergogne nel precedente *referendum* sulle trivellazioni e adesso siamo ancora di fronte a un'opinione pubblica che si vorrebbe bendare. Non lo possiamo accettare. Qui è ora di dimostrare chi è dalla parte dei cittadini e chi è dalla parte delle *lobby*.

Presidente, con questo emendamento si intende abolire l'Ordine dei giornalisti, e non siamo i

di appartenervi pone un limite a ciò che un limite non deve avere, e cioè la libertà di espressione, che peraltro nella nostra Costituzione è tutelata dall'articolo 21. Aggiunse Berlinguer che era contrario a qualsiasi requisito di titolo di studio per la professione di giornalista, trattandosi di una discriminazione assurda contraria alla libertà di stampa. Dopo questi illustri

Oggi, se vuole, è quella mattina seguente che attendeva: può dare, con il nostro voto favorevole, finalmente compimento alle sue intenzioni. Signor Presidente, un ordine a cosa serve? - a garantire ai cittadini la qualità di una prestazione e di un servizio. Ma qual è la qualità della prestazione nel giornalismo? È l'obiettività, la rispondenza dei fatti. E chi è il giudice di questo? Non certo colui che ti fa un esame a monte

che ci crediate o meno - che hanno il mandato di farci dire qualcosa che possa poi giustificare affermazioni in una determinata direzione. Accade, e ce lo vengono a dire. Allora,

sui finanziamenti e l'Ordine dei giornalisti non deve fare filtro su quello che i giornalisti scrivono. Non esiste in Francia, in Germania o in Gran Bretagna un esame di

norma, ancora una volta Matteo Renzi deve dire di fronte agli italiani - e in questo caso il Governo dovrebbe rivedere il parere negativo che ha espresso sull'emendamento - se i suoi discorsi sono cavalli di battaglia o sono cavalli di Troia *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E a voi spetta una responsabilità nel voto.

Presidente, colleghi, vi rivolgo una domanda. I quotidiani italiani sono influenzati dalle banche? Sarò ancora più preciso. «Il Messaggero» e «Il Mattino», Il Gruppo editoriale «L'Espresso» della famiglia De Benedetti, che tratta con le banche il grosso debito di un'altra società di famiglia, Sorgenia, quando di esse parla, lo fa in maniera libera o influenzata? Quale sia la risposta non uno studio pubblicato dal centro studi Stigler, dell'Università di Chicago (autore Luigi Zingales), che ha fatto un'analisi su come i giornali trattano le banche e sulle normative e le misure del Governo in questa materia. Stiamo parlando di un tema che comprende - per esempio - il decreto Bankitalia. Lo studio si è concentrato, in particolare, sull'istituzione del fondo Atlante, il cosiddetto salva banche dopo lo scandalo di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza che hanno truffato migliaia di risparmiatori, spesso anziani, povere persone, costrette - è di ieri la denuncia dell*'*Antitrust - ad acquistare azioni in cambio di un mutuo.

È stato fatto il confronto, come termine di paragone, con la stampa straniera - sul fondo Atlante hanno scritto «Bloomberg», il «Financial Times» e l'«Economist» - e quando le testate che non hanno all'estero conflitti di interessi come quelli che vi ho riportato confermano che chi è libero da questi condizionamenti scrive in maniera significativamente diversa, penso allora che vadano tolti i condizionamenti economici. *(Applausi ogni finanziamento pubblico. Non possiamo permetterci un sistema dell'informazione asservito al Governo, perché il Governo è non di tutti, ma di una parte. Rappresenta una parte, abbiamo visto anche quale parte rappresenta: lo abbiamo visto con gli emendamenti passati dalle *lobby* del petrolio sull'impianto in Basilicata e in una quantità di situazioni che ci hanno portato a chiedere le dimissioni e, in subordine, la revoca

perché noi non ci stiamo. I cittadini non ci stanno. Se andiamo a chiedere ai cittadini se vogliono che i soldi siano dati a questo tipo di

in modo equilibrato, convincente e organico. Non vi è quindi un'assoluta contrarietà nel merito della questione posta. A mio avviso, tuttavia - e mi permetta di farlo nuovamente notare

come parassiti soffocano la nostra libertà d'informazione, finalmente vengono spazzati via. Il nostro è un Paese in cui il ceto medio è scomparso

Qui dovete dimostrare coerenza, e non altrove, non sui giornali, e non come ha fatto il ministro Giannini questa mattina, quando è andata a inaugurare una scuola ad Amatrice, dimenticando che a Norcia ci sono ancora i bambini sotto le tende.

qui non si tratta di fissare per legge gli stipendi dei direttori dei giornali o degli amministratori delegati. Si tratta di dire agli imprenditori dell'informazione - lo dico non solo da parlamentare, ma anche da imprenditore che, quando si sceglie di stare sul libero mercato, non si possono chiedere i contributi pubblici. Se si chiedono i contributi pubblici, occorre stare alle regole di un'etica politica e morale, che deve prevedere un equilibrio tra le prestazioni e il riconoscimento economico delle stesse.

Pertanto, personalmente le chiedo di autorizzarmi ad apporre la mia firma a questo emendamento e mi pare di essere adeguato interprete di tutto il mio Gruppo, che le chiede anch'esso,

il relatore abbia modificato il proprio parere. Dopo le dichiarazioni e gli interventi dei due senatori che mi hanno preceduto, avrebbe dovuto essere ancor più convinto. È veramente strano che ciò che convince, guarda caso, ha creato dei dubbi nel relatore. Questa cosa non mi piace molto e non dà autorevolezza

anch'io chiedo di apporre la mia firma e quella dei senatori di Sinistra Italiana a questo suo testo, se lei permette. Poi vorrei con pacatezza cercare di far ragionare tutti quanti. La questione è molto semplice: ognuno nella propria azienda e nel proprio giornale può fare quello che vuole, anche se ci sarebbe sempre un limite in generale. Ma qui noi stiamo parlando di giornali, di testate e di società editrici che possono accedere a questo fondo, quindi stiamo parlando di denaro pubblico. a mio avviso la necessità di attenersi a delle norme, che sono quelle cui deve attenersi tutta quanta l'amministrazione pubblica; mi riferisco al limite massimo

altrettanto chiaro penso che sarebbe assolutamente opportuno e doveroso mettere un tetto alle retribuzioni.

Presidente, vorrei sottoporre al senatore Calderoli e all'Aula alcune osservazioni - che ovviamente sono, più che osservazioni, riflessioni a caldo perché non conoscevo l'emendamento e ne ho sentito parlare per la prima volta in quest'Aula quando il senatore Calderoli lo ha illustrato. Capisco che l'emendamento ha una grande efficacia comunicativa e che molte delle considerazioni che sono state svolte qui dai colleghi

il mio invito ad un attimo di riflessione. Cerco di spiegare perché ed ovviamente adopero gli strumenti che ho, che non sono strumenti squisitamente politici, ma sono anche strumenti tecnici.

ha a che fare con due principi costituzionali. Il primo principio costituzionale è quello del diritto al pluralismo nell'informazione, che però in questo caso, con questo emendamento, ovviamente deve entrare in bilanciamento con un altro principio, quello della libertà d'impresa. Ora, ciascuno di noi sa quanto pregio abbiano le osservazioni fatte dalla collega De Petris, tant'è vero che tutte le forze politiche hanno voluto inserire nel testo la condizione che le imprese che richiedono di essere ammesse alla ripartizione del fondo abbiano però nei confronti dei propri dipendenti rispettati tutti gli obblighi contrattuali e previdenziali. Ma c'è un'altra questione. Il nostro è un sistema nel quale, di volta in volta, spesso a regime e talvolta con legislazioni particolari, interi settori economici vengono ammessi al finanziamento pubblico. Nessuno ha mai chiesto che questo finanziamento pubblico fosse messo in relazione alla retribuzione corrisposta ai dirigenti di queste imprese (talvolta anche molto esuberanti, ovviamente,

tutta una serie di questioni e di vertenze aventi ad oggetto il fatto che vi siano imprese operanti nel libero mercato ammesse a un finanziamento pubblico, purtroppo spesso più cospicuo di quello che verrà assicurato dalla ripartizione del fondo, e che non sono tenute ad osservare nessun limite nella retribuzione Detto questo, mi permetto di chiedere all'Aula una pausa di riflessione sulla decisione, che potrà avere due forme. La prima è quella che opportunamente il Governo ha rappresentato: quella di presentare un ordine del giorno impegnandoci a ragionare su questo tema. Nel caso questa forma non venga accolta dall'Aula, in quanto non ritenuta soddisfacente, quella di fermarci nella riflessione su questo emendamento, che possiamo anche affrontare, dal momento che non sussistono problemi di preclusione, successivamente.

Io posso concordare sui principi enunciati dalla presidente Finocchiaro rispetto alla libertà di informazione. Ma noi abbiamo già previsto casi di esclusione rispetto alla possibilità di percepire i contributi. Abbiamo escluso gli organi di informazione dei partiti che comunque godono della libertà di informazione - e dei movimenti sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Siamo andati quindi ad escludere una parte che, comunque, rientra nella libertà dell'informazione. Abbiamo escluso tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati in mercati regolamentati e anche questi rientrano della libertà dell'informazione. Quindi, prevedere un ulteriore requisito rispetto al fatto che si possa accedere o meno a questi contributi non introduce un nuovo principio, ma introduce un altro criterio. Adesso, non parlando in termini giuridici, ma molto fuori dai denti, tutti i settori dell'editoria, soprattutto a livello dell'emittenza locale, vivranno o decederanno sulla base dei contributi che riceveranno. Credo sia sacrosanto un sostegno alla libertà dell'informazione.

bisogna disciplinarlo meglio, non ci sono santi, noi non andiamo a toccare i tetti retributivi degli amministratori e direttori di giornali. che se tu vuoi vivere con i soldi che ti dà anche lo Stato tu al tuo direttore più di 240.000 euro non gli puoi dare. A me sembra una cosa sacrosanta ed anche equa e credo che l'Aula la approverà, visto che alla fine mi sembra che sia il Governo che il relatore si rimettano all'Aula. Mi dispiace che il relatore abbia modificato la propria posizione anche per il carico politico. Qui non c'è un carico politico, qui c'è solo il buonsenso: vi diamo dei soldi, non buttateli via.

a lungo in Italia di tante aziende importanti, anche private, che hanno ricevuto sostegni pubblici sotto varie forme, ammortizzatori sociali e quant'altro. Poi alcune portano la sede

Si potrebbe anche parlare di Ryanair. Il Governo recentemente si è vantato di un accordo con Ryanair che fa volare a poco prezzo però poi bisognerebbe conoscere i contratti di lavoro dei dipendenti, i soldi che prendono dagli aeroporti, cioè dalle ex Province e dalle città.

*manager* o direttori che guadagnano più di 240.000 euro. Quindi è un principio, non è una norma *ad personam*, o *ad personas*,

posta, telefono ed eventuali tariffe agevolate perché qualcosina, secondo me, ancora c'è anche nel settore non direttamente sussidiato anche se quelle sono condizioni di vantaggio rispetto al alcune tariffe.

generoso. Lo dico anche a noi stessi. Qui si parla tanto delle caste, della casta, dei trattamenti dei parlamentari e quant'altro che giustamente vanno rivisti, in parte sono già stati rivisti e forse non sarà abbastanza, ma qui parliamo di cifre che sono letteralmente al di sopra del trattamento massimo della presunta casta. perché non si deve approvare questa norma? La trovo assolutamente logica, di buonsenso: non nega il diritto a fruire di sussidi pubblici, ma prevede che queste

sul mercato, hanno dei sussidi; ne parleremo quando ci arriveremo. Lo Stato ha anche un dovere, a volte; gli ammortizzatori sociali sono una cosa utile: quante crisi risolvono e affrontano? Poi, se chi ne fruisce ha una condotta un po' più austera, tutto sommato si fa anche un lavoro corretto nei confronti della comunità che soccorre chi è in crisi, ma che ottiene in cambio un comportamento più virtuoso. Lo ricordo a noi stessi, che siamo giustamente al centro dell'attenzione e non si capisce perché dobbiamo avere una immotivata generosità a beneficio di terzi, che francamente possono vivere lo stesso, anche con quel tetto. La mia, quindi, è un'adesione non polemica ma di buonsenso, che mi auguro sia ampiamente condivisa dall'Assemblea del Senato.

rispondesse alla finalità suprema e superiore che ci vede impegnati molto spesso a commentare e illustrare i testi degli emendamenti che proponiamo, ossia migliorare la qualità della produzione legislativa. La collega Finocchiaro, con la sua consueta prudenza e con la riconosciuta competenza, ha riconosciuto che l'emendamento non era stato approfondito in modo adeguato e quindi, sostanzialmente, ha esposto il suo pensiero, offrendo anche delle valutazioni in ordine alle ipotesi di rischio, tutte - mi pare - connesse all'eventualità che l'approvazione di questo emendamento possa avere delle ricadute negative, determinate dall'ipotetica estensione del provvedimento stesso a una fattispecie che superi quella che si intende normare. Prima il collega Candiani, poi lo stesso proponente, senatore Calderoli, in modo puntuale e preciso, con l'aggiunta delle osservazioni fatte dal collega Gasparri, credo però abbiano aggiunto elementi valutativi ed esplicativi sufficientemente chiari che, anche a me che avevo approfondito in modo assolutamente insufficiente il testo dell'emendamento, hanno portato a formare un solido convincimento che si tratti di una proposta emendativa da sostenere. Ho troppa stima del collega Cociancich per ritenere che la modifica del suo parere positivo

che, anche attraverso gli interventi che abbiamo ascoltato, che sono di pregio e convincenti nel merito, si possa superare il sospetto che il Governo induca induca la maggioranza dell'Assemblea ad esprimersi in un modo funzionale alla volontà del potere costituito. Il potere costituito è quello che si forma attraverso la maggioranza che esprimerà

l'approvazione di un ordine del giorno con cui il Governo si impegna ad affrontare il tema ovvero l'accantonamento. allora spontanea la domanda: se la norma, così come è stata immaginata dal senatore Calderoli, presenta dei vizi di incostituzionalità

chiedere un impegno del Governo ad approvare e ad affrontare il tema sempre sulla base di un principio incostituzionale? Se vi sono dei vizi di incostituzionalità nella previsione normativa del senatore Calderoli, vi sono sia nell'emendamento che andiamo ad approvare sia nell'eventuale ordine del giorno. Non si comprende come si possano ritenere non superabili questi rilievi di incostituzionalità

anche tecnico visto che talvolta le questioni vengono opportunamente poste sul piano tecnico. Se ci dobbiamo confrontare anche sul piano tecnico, non vi sono problemi e possiamo farlo. e possiamo farlo. Sul piano tecnico ribadisco che non ritengo vi sia alcun profilo di incostituzionalità della previsione normativa

entrata in campo anche la Presidente della Commissione suggerendo l'accantonamento. Ora questa posizione viene anche assunta dal relatore. Questo emendamento è datato agosto 2016: non è arrivato oggi in Assemblea, ma risale al periodo della chiusura dei nostri lavori, quando ci siamo dedicati ad altri provvedimenti dopo quello in discussione. So benissimo come funziona il "giro del fumo":

Volete fare in modo che le risorse pubbliche vengano utilizzate nella più libera discrezionalità da parte di questi soggetti, io credo che questo sia ingiusto. Sull'accantonamento decide il Presidente, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, quindi sarà una sua spettanza.

di essere disponibili a pagare quelle cifre a coloro che prendono i soldi non nostri, ma dei contribuenti, allora, ragazzi miei, la mia posizione cambia rispetto a tutto il resto del provvedimento sia sia nel senso del voto finale sia nel comportamento in Aula, perché a tutto c'è un limite, anche al buon senso e alla decenza. Non facciamo più dei provvedimenti che risultino a tutti gli effetti come delle marchette.

e per l'innovazione nell'informazione. Riserviamo queste risorse alle società composte prevalentemente da giornalisti e che utilizzano prevalentemente l'assunzione in forma stabile. Sappiamo qual è la pratica di sfruttamento capillare e pesantissima del lavoro dei giornalisti che vengono pagati a cottimo (c'è ancora il cottimo nel giornalismo), con retribuzioni incompatibili con la qualità della scrittura e l'analisi attenta dei fatti. I giornalisti, a volte, possono anche essere indotti in errore dal modo in cui vengono retribuiti e sono costretti a lavorare. Questo dimostra una cosa su tutte, ossia che il Movimento 5 Stelle non è contro il giornalismo o contro i giornalisti; semmai è contrario a un sistema dell'editoria che è profondamente malato ed è malato dall'alto nel momento in cui la politica lo occupa malamente. Noi chiediamo semplicemente questo: che ci sia una rispondenza effettiva tra la finalità dichiarata nella legge e come vengono utilizzati i finanziamenti.

Non sembra una cosa congrua - in un ambito dove si cerca di incoraggiare alla programmazione, all'innovazione e così via - garantire questi finanziamenti, sia pure in modo limitato, per un periodo a sua volta limitato. Meglio, quindi, cinque anni che tre, ma resta in sé una limitazione difficile

Qui sono comprese le fondazioni riferibili a soggetti politici, singoli esponenti, partiti, correnti, e se la norma esplicitamente, cioè dalla porta, esclude i partiti e i sindacati, non vogliamo che questi soggetti vengano riportati dentro dalla finestra, magari in maniera

Presidente, abbiamo diversi esempi di testate giornalistiche riferite direttamente o indirettamente a partiti o ad esponenti politici:

non ci deve essere collegamento diretto, non ci deve essere nemmeno collegamento indiretto. La politica deve stare fuori dall'editoria, se non altro deve star fuori dai contributi all'editoria e in questa sede dobbiamo dire in maniera chiara e trasparente se vogliamo continuare a elargire sotto banco finanziamenti a questi organi, oppure se devono essere esclusi. Tra l'altro, quando questi fanno riferimento al partito del presidente che si tratti ancora dello stesso partito, visto che a volte viene il dubbio), dovremmo ricordarci che lui si era dichiarato contrario a questi finanziamenti mentre ora si sta cambiando rotta. Noi siamo coerenti su questo; abbiamo proposto emendamenti soppressivi *tout court* del finanziamento e vorremmo che, almeno negli aspetti di dettaglio, fosse riconosciuto che ci stiamo sforzando in tutti i modi di introdurre misure, anche le più

dal mondo dell'informazione.

Presidente, conosciamo tutti quella citazione per cui il giornalismo, l'informazione, è dire qualcosa che qualcuno vuole che non si sappia; tutto il resto è propaganda. di porre un limite alla raccolta pubblicitaria da parte delle testate, perché se un giornale viene finanziato per più del 30 per cento dei suoi costi complessivi dalla pubblicità, è lecito dubitare se faccia informazione o *réclame*. Ciò detto, la raccolta pubblicitaria doveva essere il vero cuore del pluralismo, perché ad esempio noi sappiamo quanto sia ingessato il sistema dell'emittenza per il fatto che pochissime agenzie di pubblicità

giornalisti e direttori dalle reti pubbliche ci sta a dire che andiamo sempre più verso un sistema dell'informazione

estremamente "mirata", perché va a colpire il problema e propone una soluzione che realizza immediatamente una redistribuzione delle risorse tra tutte le testate, mettendole tutte su un piano di parità. Proprio questa parità era tra i principi

Quando diciamo di escludere dai finanziamenti le imprese «che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso»

Presidente, tra le cause dell'emergenza spazzatura ci sono i giornali; non i giornali intesi come testate, ma quelli che vengono stampati perché il sistema dei contributi e delle sovvenzioni è drogato ed è tarato sulle copie distribuite anziché sulle copie vendute.

usiamo risorse pubbliche per sprecare risorse materiali. A tutto questo si può porre rimedio votando questo emendamento, che prevede che il contributo debba essere elargito in base alle

il senatore che è intervenuto per ultimo mi ha fatto venire alla mente quando - lo ricorderà il senatore Casini - fui liquidatore della testata "La Discussione", che quindi ho amministrato per un certo periodo. Ebbene, si verificava esattamente proprio quello

facevano sì che si stampassero più copie rispetto a quelle che poi venivano vendute. È un fatto antico, che si verifica da tempo; è sempre stato così. Se l'emendamento del senatore del Movimento 5 Stelle mira ad evitare questo sconcio che dura da anni e che io ho potuto verificare personalmente sotto il profilo professionale, ebbene non posso

Essa prevede che, quando un soggetto, per ottenere il contributo, rilascia dichiarazioni mendaci, egli sia punito

si sono avute, sebbene si sia reagito con grande prontezza. Io mi permetto di ricordare qui un lavoro che è stato, secondo me, prezioso, perché a causa del terremoto

protezione animali è stato attivo con la Protezione civile già dalla mattina del 24 agosto. Ha svolto una prima fase di lavoro e poi una seconda fase. Ci sono stati interventi su più di 950 animali. È stato fatto un lavoro prezioso sia nei confronti di animali da affezione (più di 300 cani e più di 200 gatti), sia degli animali da reddito (quasi 400); 400); esseri senzienti essenziali alla vita e all'affetto delle persone con le quali avevano fino a quel momento vissuto. vissuto. Tutti abbiamo potuto apprezzare i momenti di grande emozione che hanno visto il ricongiungimento di animali con l'unico rappresentante umano ancora presente della loro famiglia e penso che quel valore di affinità sia un altro grande regalo che il nostro mondo ha saputo esprimere. Deve essere riconosciuto all'ENPA questo impegno, con 41 persone e con i tanti mezzi

Certo, i ricongiungimenti non sono stati tutti quelli possibili: su 300 cani solo 4 erano dotati di *chip*. Vuol dire che l'impegno del nostro Ministero della salute deve essere molto più forte nella lotta al randagismo. Un impegno più forte significa dare risorse alle ASL e alle Regioni per poter fare progetti mirati

di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», premesso